Resta confermato che questa settimana è essenzialmente dedicata al seguito del disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario. La conclusione del provvedimento è stata concordemente prevista per la giornata di venerdì 13 o, se necessario, nella seduta antimeridiana di sabato 14 luglio. La Presidenza si farà garante, nell'esercizio dei propri poteri, del rispetto di quanto unanimemente stabilito. La seduta pomeridiana di oggi si concluderà alle ore 20, anziché alle ore su richiesta del Governo. Giovedì 12 luglio, alle ore 12, è convocato il Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale (settimo scrutinio a maggioranza dei tre quinti dei componenti). Voteranno per primi i deputati. La chiama dei senatori inizierà intorno le ore 13,45. È stato pertanto anticipato di un quarto d'ora l'orario di chiusura della seduta antimeridiana del Senato. Restano compresi nel calendario della settimana - se l'andamento dei lavori lo consentirà - il seguito del disegno di legge recante norme fiscali e l'avvio della discussione generale del decreto-legge in materia di energia. La discussione generale avrà comunque inizio, anche con un eventuale voto di questioni incidentali, nella seduta antimeridiana di martedì 17 luglio. In apertura della seduta pomeridiana del 17 luglio, saranno poste ai voti le dimissioni presentate dal senatore Selva. Il calendario della settimana prossima prevede poi il seguito del decreto-legge in materia di energia, l'eventuale seguito del disegno di legge recante norme fiscali, il seguito della legge comunitaria e, ove concluso dalla Commissione competente, l'esame del disegno di legge di riforma del sistema di informazione e sicurezza. Per quanto riguarda il documento presentato dal senatore Calderoli al fine di richiedere comunicazioni del Governo sullo stato delle missioni internazionali, il Presidente, sentito il Governo, proporrà ai Capigruppo la data di un prossimo dibattito. Infine, la Conferenza dei Capigruppo ha concordato in linea di massima, anche in relazione al calendario della Camera dei deputati, la data di conclusione dei lavori dell'Assemblea prima della pausa estiva intorno al 2 agosto. Nelle prossime riunioni della Conferenza saranno definiti i provvedimenti prioritari da inserire nel calendario prima di tale data, fermo restando che il Documento di programmazione economico-finanziaria potrà essere esaminato a partire dalla giornata di mercoledì 25 luglio.

si sono registrati notevoli disservizi sul *server* delle Agenzie delle entrate ed i commercialisti, che si fanno carico di questi adempimenti, erano nell'impossibilità di procedere ai collegamenti per tali gravi disfunzioni. Ora, tutto ciò determina gravi conseguenze sul piano delle sanzioni rispetto al pagamento delle obbligazioni tributarie; si tratta di intervenire in maniera corretta, tenendo conto di questo stato di difficoltà,

intervengo solo per comunicare che, a norma dell'articolo 79 del Regolamento, il Gruppo Insieme con l'Unione-Verdi-Comunisti Italiani fa proprio il disegno di legge n. 1396

in Italia. I NAS hanno sequestrato, in varie aziende che vendono prodotti, circa 20.000 tubetti di dentifricio Colgate prodotto in Cina ed abusivamente entrato in territorio italiano. In Spagna sono stati sequestrati 100.000 di questi tubetti di dentifricio, contenenti sostanze che, da un esame

sta riportando alcune notizie relative al voto degli italiani all'estero riguardante il Senato della Repubblica:

mettere a disposizione della Commissione di merito o se si ritenga di fare qualche passo per cercare di acclarare la verità. Infatti, non possiamo restare nel sospetto che la composizione di quest'Aula sia il frutto di un broglio elettorale.

Non ho ancora avuto segnalazioni o richieste, ma naturalmente, se ci saranno, ci premureremo, come Presidenza, di fornire tutti gli elementi alla Giunta delle elezioni per consentire un approfondimento

Credo che tutti i Gruppi siano rimasti fermi nelle loro posizioni e che queste posizioni ben si rappresentano, specialmente per il centro-destra, negli emendamenti presentati al testo oggi in esame. Io credo che questa maggioranza abbia voluto correggere gli eccessi della riforma Castelli e comunque abbia voluto

e quindi non ci spaventa il fatto che oggi, contro questa riforma, manifestino sia gli avvocati sia l'Associazione nazionale magistrati, la quale sembra sia in procinto di proclamare uno sciopero.

tendevano alla separazione delle carriere, i magistrati tendono a rimanere nel loro ufficio, per quanto è possibile rimanerci, pur mutando funzione. Queste due contrapposizioni, che - ripeto - sono speculari tra loro, urtano contro la sensibilità dei cittadini, che invece vorrebbero una magistratura che appaia anche all'esterno divisa per funzioni, per quello che la Costituzione prevede: un magistrato che non si presenti un giorno in veste di accusatore e il giorno dopo seduto sullo scranno del giudice. Così pure gli avvocati dovrebbero capire che i magistrati vanno divisi per funzioni, non per carriere, che la carriera unica, tutto sommato, li accomuna in una cultura della giurisdizione.

nel modo in cui è scritto nel testo che presentiamo oggi e che credo sia la posizione più avanzata ed equilibrata che la maggioranza poteva raggiungere. Quindi, spero che il prosieguo della discussione e delle votazioni sia sereno e che alla fine si possa dare un giudizio positivo sul lavoro ottimo che la Commissione ha svolto,

che hanno mostrato grande senso delle istituzioni e che non hanno minimamente fatto ricorso all'ostruzionismo, e infine

sento il dovere di iniziare la mia replica esprimendo un convinto e non rituale omaggio al Parlamento, anche in questa occasione luogo essenziale di confronto democratico, massima espressione di sovranità popolare, nel quale la volontà dei cittadini viene trasfusa in provvedimenti che regoleranno per il futuro la vita del Paese. Come sapete, onorevoli senatori, il provvedimento oggi in esame costituisce l'epilogo di una lunga e complessa vicenda da ultimo segnata dalla legge con la quale l'ottobre scorso venne sospeso il decreto legislativo concernente l'accesso e la carriera dei magistrati emanato dal precedente Governo. Avevamo ritenuto in quel momento assolutamente necessario provvedere alla modifica di quel testo, che a nostro avviso si poneva in contraddizione con l'esigenza di modernizzare e rendere più funzionale la giustizia del nostro Paese, nel pieno rispetto, però, dei fondamentali principi costituzionali. Il testo approvato alla Commissione giustizia, pur se migliorabile ed emendabile in alcuni suoi punti (e su questo esprimo la disponibilità del Governo, specie se questi punti sono utili per eliminare negative ruggini ideologiche dal dibattito sulla distinzione delle funzioni dei magistrati),

un punto di equilibrio, che ritengo virtuoso, tra le diverse sensibilità esistenti nel mondo della giustizia e nell'intero Paese, che trovano proprio nel Parlamento e non altrove la loro compiuta espressione. Il rapporto dialettico tra maggioranza e opposizione, e quello pure esistito - perché non riconoscerlo? - all'interno della mia stessa maggioranza, realizzano in questo quadro il loro alto valore di attuazione del metodo democratico posto a fondamento della vita repubblicana. Immiserire la fibra costitutiva delle nostre istituzioni sulla base di ripensamenti postumi mi sembra appartenga più alla sfera delle ripicche vanitose o dei calcoli politici di breve respiro piuttosto che all'ambito, quanto mai necessario in una materia come la giustizia, della doverosa attenzione dell'intero Parlamento agli interessi di lungo periodo del nostro Paese. interessi certo troverebbero un quadro favorevole alla loro soddisfazione laddove si riuscisse (questo è stato il tentativo in parte riuscito e spero possa riuscire nel corso del dibattito) a far superare la stagione delle guerre puniche fra mondo politico e magistratura.

Autonomia e indipendenza della magistratura sono in questo contesto - voglio dirlo con assoluta chiarezza e fermissima convinzione - valori irrinunciabili. Ma l'autonomia non deve essere soffocata dalla tentazione di quei magistrati all'autoreferenzialità, così come è estraneo all'idea stessa di democrazia che un valore così alto e fondante possa essere difeso da qualcuno in particolare, laddove la sua assoluta garanzia si trova non in qualcuno di noi, ma nella Costituzione repubblicana. repubblicana. Anche rispetto a questo provvedimento, non ci sono finti pretoriani che, con pensiero postumo e debole, possano ergersi ad esclusivi Don Chisciotte della legalità. Prima di una rapidissima analisi di alcuni punti qualificanti del testo oggi proposto al vostro esame, permettetemi un'altra considerazione. la giustizia abbia bisogno di valori e princìpi alti, non di sterili contrapposizioni ideologiche. Essa ha bisogno di modernizzazione ed efficienza, perché è fattore imprescindibile di progresso civile e di crescita economica del Paese. Oggi la SVIMEZ annuncia che assieme a questa drammatica emigrazione di ritorno dal Mezzogiorno, rispetto al Nord del Paese, uno degli aspetti che più incide in negativo sullo sviluppo del Mezzogiorno è dato dalla giustizia civile, più lenta nella sua progressione per quanto riguarda il Nord del Paese. Una giustizia inefficiente è una giustizia non credibile e, al termine di questa giustizia non credibile e di questa non credibilità, ciascuno degli attori del processo (e mi riferisco agli avvocati, ai magistrati, al personale amministrativo, ai cittadini) ne sopporterà i costi in termini di mancanza di legittimazione, perché non c'è sottesa, rispetto a questa giustizia, l'anima da parte della popolazione. Un ordinamento giudiziario moderno e rinnovato costituisce il fondamento di una giustizia capace di assumere pienamente l'alto compito che le è proprio. Esso deve essere aperto agli apporti esterni alla magistratura e, al tempo stesso, garante delle prerogative costituzionali ad essa spettanti a tutela dei cittadini e dei loro diritti; fattore di sviluppo e di riconoscimento della professionalità e della responsabilità necessaria per l'esercizio delle funzioni giudiziarie; strumento al tempo stesso di selezione trasparente dell'uomo giusto - si spera - nel posto giusto; elemento di garanzia della terzietà e dell'imparzialità del giudice. Questo tipo di ordinamento che vi è stato proposto, onorevoli senatori, ritengo che possiamo costruirlo assieme, come in realtà si è convenuto e come è capitato ed è avvenuto finora, nel lungo periodo e al di là delle contingenze politiche particolari. Questa essenziale componente e l'apparato istituzionale hanno bisogno dell'apporto calorico e dell'energia di tutti quelli che sono qui e devono essere protagonisti parlamentari. Passo ora a scattare qualche fotografia nel dettaglio del paesaggio, così come è stato confezionato. Per l'accesso in magistratura si è conservato il modello di concorso di secondo grado verso cui già si orientava la precedente riforma. Crediamo di aver migliorato quel meccanismo, prevedendo che possano partecipare alle prove non i semplici laureati in legge, ma coloro che abbiano già acquisito titoli ulteriori particolarmente significativi. Si tratta, dunque, di una platea di aspiranti ben qualificata per esperienza di settore, per capacità scientifica, per cultura, il che garantisce a priori la possibilità di una seria selezione. È stata poi conservata, all'interno di questo contesto e di questo segmento particolare, la soppressione di quel riscontro psico-attitudinale previsto dalla cosiddetta riforma Castelli, che tante perplessità, per la verità, aveva suscitato anche in sede scientifica, così come eliminata risulta l'obbligatoria anticipata opzione tra funzioni giudicanti e funzioni requirenti. Le altre modifiche al sistema di accesso riguardano la formazione delle commissioni esaminatrici, lo svolgimento dell'attività valutativa, la definizione anticipata dei criteri per la valutazione omogenea degli elaborati, la distinzione in gruppi di lavoro nella prospettiva di accelerare l'*iter* dei concorsi in modo che si possa rispettarne la cadenza annuale. Non guerre puniche, dunque, ma laica ricerca di efficienza e anche di condivisione. Anche le modifiche apportate alla Scuola superiore della magistratura sono state finalizzate a garantirne la funzionalità operativa, con alcune semplificazioni organizzative dovute alla necessità soprattutto di comprimerne i costi. In Commissione - ne do atto al relatore e al presidente Salvi, ma all'intera Commissione, per la verità - si è trovato un opportuno contemperamento tra le esigenze di autonomia del nuovo ente e la esigenza che i bisogni formativi dei magistrati siano correttamente individuati e al tempo stesso soddisfatti. La nuova disciplina che ne deriva è tale da accentuare l'autonomia scientifica, didattica e gestionale della scuola, esaltandone l'apporto alla preparazione dei magistrati di prima nomina, alla formazione permanente e di riconversione, alla creazione di una vera e propria cultura manageriale dei capi degli uffici, perché anche di questo si tratta: realizzare una sorta di nuova cultura dell'organizzazione all'interno della struttura giudiziaria. L'attuale composizione del consiglio direttivo della Scuola, che unisce alla magistratura anche la competenza e la professionalità dell'università e dell'avvocatura, è tale da assicurare la presenza di professionalità idonee a consentire il perseguimento dei fini sicuramente molto ambiziosi - e giustamente ambiziosi - che la Scuola intende perseguire. Sono personalmente persuaso che la formazione professionale dei magistrati rappresenti un fattore cruciale di positiva innovazione del sistema giustizia e, al tempo stesso, di salvaguardia dell'autonomia e dell'indipendenza della stessa magistratura. Tale duplice natura della formazione trova del resto precisa risonanza costituzionale negli articoli 105 e 110 della nostra Carta fondamentale. In tali disposizioni, il rapporto potenzialmente dialettico tra autonomia e indipendenza di ogni magistrato, la cui tutela è fondamentalmente affidata al Consiglio superiore della magistratura, e interesse pubblico alla corretta organizzazione e al buon funzionamento dell'amministrazione della giustizia, responsabilità primaria del Ministro, rendono costituzionalmente necessitato il metodo di leale e piena collaborazione tra poteri dello Stato. La Corte costituzionale ha più volte negato che potesse essere tracciata, sulla sola base dell'articolo 105 della Costituzione, una netta separazione di compiti tra Ministro e Consiglio superiore della magistratura. È a tale vincolo di metodo nei rapporti tra CSM e Ministro, animati per la verità dal comune impegno e dal confronto aperto e costruttivo e - per utilizzare le stesse parole della Corte costituzionale - «realmente orientati al superiore interesse pubblico di operare (...) le scelte più idonee», che ho cercato e abbiamo cercato di attenerci nel disegnare la struttura e i compiti della Scuola, assicurando la partecipazione di entrambi gli organi interessati e ritenendo ineludibile la pratica dell'intesa e della collaborazione. Del resto, le esigenze di efficienza e buon andamento dell'amministrazione della giustizia rafforzano il fondamento costituzionale della partecipazione del Guardasigilli alle decisioni sulla formazione, individuando nell'articolo 97 della Costituzione il necessario riferimento dei poteri riconosciuti nell'articolo 110. Tanto più che l'efficienza del servizio giustizia postula l'apporto di tutti gli operatori giuridici ed il coinvolgimento della comunità scientifica, allorché la Scuola, sebbene esclusivamente riferita alla magistratura nella sua denominazione, è chiamata ad offrire i suoi servizi all'intero sistema giustizia, coinvolgendo cioè nella formazione, quali utenti non secondari, oltre che i magistrati onorari, anche gli operatori della giustizia e gli iscritti alle scuole di specializzazione forense. Anche in questo specifico settore si è tenuto conto delle osservazioni provenienti dalle istituzioni, anche dal CSM e dal mondo giudiziario e forense, cercando così di assicurare una sintesi positiva e orientata a quello che viene chiamato l'interesse generale. Ho quindi proposto e condiviso l'iniziativa di modifica dell'originario testo del disegno di legge del Governo riguardante la composizione del comitato direttivo della Scuola,

Per quanto riguarda i consigli giudiziari, su cui molto si è discusso, le uniche divergenze di opinioni che si sono riscontrate, sia in Commissione che in Aula, concernono, per la verità, la mancata inclusione tra i compiti affidati ai componenti estranei alla magistratura, dell'attività di valutazione dei magistrati.

debbo dire che la scelta operata dal Governo, prima, e dalla Commissione, poi, è stata nel senso di non prevedere la partecipazione degli avvocati alla valutazione dei magistrati, pur essendo in verità confermato il loro coinvolgimento nelle scelte attinenti all'organizzazione degli uffici giudiziari e le modalità di messa a disposizione dei relativi servizi. Devo ricordare a quanti magari possono almanaccare in maniera differente da questa impostazione, che nel progetto licenziato dalla precedente maggioranza il compito di valutare i magistrati non era stato attribuito ai membri non magistrati dei consigli giudiziari. Appare quindi scarsamente comprensibile, per la verità, l'accusa che vedo rivolta in qualche circostanza, che fa capolino ogni tanto, per cui l'attuale maggioranza avrebbe scelto in maniera diversa: in realtà, siamo nella traiettoria, nel cono d'ombra di quanto è stato scelto anche precedentemente dalla vecchia maggioranza. Ma debbo dire che non è questo l'aspetto più importante della vicenda. Il vero nodo della questione consiste nel valutare se la partecipazione degli avvocati nelle valutazioni della professionalità dei magistrati assolutamente - necessaria per assicurare il miglior funzionamento del sistema. In realtà, in questo caso non mi sembra che possa essere così, dal momento che il procedimento di valutazione della professionalità viene ora strutturato in modo da garantire che i consigli giudiziari operino una valutazione preliminare dei magistrati sulla base di una gran quantità di riscontri ed elementi effettivamente concreti. Tra di essi figurano anche le informazioni e le segnalazioni trasmesse dai consigli degli ordini degli avvocati, quindi non c'è una reticenza rispetto a quale possa essere il giudizio emesso da parte dei consigli degli ordini degli avvocati. che il compito di valutare la professionalità del magistrato è riservato al solo Consiglio superiore della magistratura, rispetto al quale l'attività del consiglio giudiziario si atteggia unicamente quale attività istruttoria preliminare. Al parere del consiglio giudiziario devono essere allegati tutti gli elementi presi in considerazione, determinati secondo parametri assai stringenti, ivi comprese le informazioni ed osservazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati. La soluzione prescelta consente quindi di considerare le osservazioni degli organi istituzionali dell'avvocatura, evitando al contempo il prodursi di problematiche, anche in ambito processuale, da più parti segnalate. Interventi più consistenti sono stati invece necessari in relazione a quella parte del decreto-legislativo n. 160 del 2006 in tema di progressione di carriera. Ciò perché al farraginoso sistema concorsuale

Come ho detto in sede di presentazione del mio programma dinanzi alle Commissioni giustizia delle due Camere, il sistema concorsuale del decreto a parte lo stigma impiegatizio che sembrava riprodurre l'ordinamento del 1941, poneva per la verità serie perplessità dal punto di vista della mera funzionalità. Quanto volte e per quanto tempo ogni magistrato si sarebbe sottratto all'ordinario esercizio della sua attività per dedicarsi esclusivamente alla preparazione dei vari concorsi interni? Come avrebbe potuto non distrarre il suo impegno dalla giurisdizione? Quale stimolo ad un carrierismo indifferente alle sorti della giustizia un simile sistema avrebbe inoculato nell'ordine giudiziario? In sostanza, la possibilità di partecipare ai concorsi, con la prospettiva di vantaggi di carriera e i relativi risvolti economici, avrebbe potuto indurre molti a scegliere questa strada, abbandonando quegli uffici di primo grado dove si adottano le decisioni con il maggior impatto sociale, con la maggior rilevanza sociale. Tutto ciò in contrasto in contrasto con l'interesse e con il primato del cittadino a rivendicare un magistrato esperto fin dal primo grado di giudizio del processo. Viceversa, le valutazioni periodiche a tempi ravvicinati costituiscono non solo il presupposto per altre funzioni, ma anche importanti momenti di verifica suscettibili di concludersi, se di esito negativo, con il blocco della progressione economica o con la destinazione ad altra funzione di chi si riveli inidoneo, o con la rimozione dei magistrati che non superino successive valutazioni di merito. Sul punto, vale la pena di segnalare che questo tipo di previsione costituisce un *unicum* in tutto il pubblico impiego, non essendovi (di qua la specificità) altri esempi di valutazioni così ravvicinate nel tempo che si estendano per tutto il periodo di attività lavorativa e che si possano concludere con una valutazione che comporti la risoluzione del rapporto di lavoro stesso. Tali verifiche si fondano sulla raccolta e sull'esame di tutti gli elementi idonei a ricostruire l'attività di ciascun magistrato, sulla base di criteri oggettivi previsti dal Consiglio superiore della magistratura e dei rapporti dei capi degli uffici. In definitiva, siamo in presenza di un sistema di valutazione insieme rigoroso, efficiente e rispettoso di uno *status* che non deve assumere l'idea del privilegio come tale, ma deve essere garanzia del buon esercizio della giurisdizione al servizio del cittadino. Quanto alle funzioni di legittimità, a differenza dell'ordinamento Castelli, è stato garantito che, in linea con la Costituzione, il sistema resti nell'ambito della competenza del Consiglio superiore. Tuttavia quest'ultimo si avvarrà di un apposito gruppo di magistrati, professori universitari e avvocati per la valutazione dei provvedimenti degli aspiranti finalizzata al riscontro delle specifiche e proprie attitudini. Insomma, per l'accesso alle funzioni di legittimità la prospettiva è diversa: un magistrato, per quanto bravo nell'attività di merito, può non essere in grado di svolgere una funzione di legittimità e perciò l'aspirante deve saper dimostrare la capacità di analisi delle norme, ove l'indagine sulla identità normativa è cosa ben diversa dalla ricostruzione del fatto, sia pure *sub specie iuris*. È stata poi introdotta, onorevoli senatori, la possibilità, per i magistrati che abbiano conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità, di partecipare ad una procedura riservata in relazione al conferimento del 10 per cento dei posti vacanti in Cassazione, qualora siano in possesso di titoli e capacità che li rendano comunque idonei alla funzione. Detta anticipazione del conferimento delle funzioni di legittimità presso la Corte non comporta, però, alcuna conseguenza, né sul piano giuridico né su quello economico, evitando in questo modo le distorsioni insite in sistemi acceleratori della progressione economica stessa. Dinamizzare e anticipare l'accesso all'esercizio delle funzioni di legittimità appare, in questo quadro, assai utile e non foriero di rischi per il complessivo assetto della magistratura italiana. Su questi presupposti di controllata idoneità e sulla base di rigorose procedure concorsuali per titoli, nonché di partecipazione a specifici corsi, si realizza l'attribuzione di incarichi semidirettivi, direttivi ed apicali. In proposito, si deve tener conto anche delle specifiche attitudini organizzative e di gestione e della capacità di rapporto con il personale e l'utenza (la scuola, da questo punto di vista, ha uno specifico settore di formazione), nella prospettiva, sottesa all'articolo 107 della Costituzione, di porre davvero l'uomo giusto al posto giusto (così si spera). Un'altra questione sulla quale vi è stata una forte contrapposizione - diciamo la verità - è costituita dalle modalità del passaggio dalla requirente alla giudicante e viceversa. Il passaggio, nella formulazione della Commissione, è consentito a seguito della frequenza di un corso di qualificazione professionale è subordinato allo svolgimento delle medesime funzioni per almeno cinque anni e ad un giudizio di idoneità specifica per il quale è possibileacquisire il parere del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati; tale passaggio non è possibile però in una sede compresa nella medesima Regione, nel capoluogo del distretto determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, e, comunque, per un numero di volte superiore a quattro nel corso dell'intera attività di servizio. sul punto si è comunque aperti a soluzioni migliorative (laddove ci fosse questa possibilità od opportunità), che venissero presentate nel corso della discussione dai colleghi senatori. Quello però che va evitato è il sovraccarico ideologico di una disputa, che può e deve trovare una soluzione non traumatica, ma utile ed idonea, cui ha fatto cenno anche il relatore in premessa del suo intervento. Vorrei a tal proposito sottolineare come quella separazione delle carriere, che ancora oggi molti, nel mondo politico e nell'avvocatura, propugnano, oltre agli ostacoli di ordine costituzionale, a norma di Costituzione vigente, che ne impediscono la realizzazione per legge ordinaria, non è stata prefigrata neppure nella scorsa legislatura in un quadro dotato, dal punto di vista dell'impianto parlamentare, di ben altra attrezzatura per quanto riguarda i numeri da parte della maggioranza. Riproporla oggi surrettiziamente mi sembra francamente un calcolo politico che non è giusto riportare in questa questione che, comunque, ha un valore di natura istituzionale. Non può, infine, sottacersi l'importanza dell'introduzione del principio di temporaneità di tutte le funzioni direttive e semidirettive; innovazione che comporta, come corollario, un sistema di conferimento degli incarichi basato su concorsi finalizzati ad assicurare che la scelta cada su candidati individuati solo per le loro capacità. Una questione separata costituiscono le norme che sono state oggetto della proposta di stralcio da parte della Commissione che le ha ritenute, per la loro non diretta correlazione con il decreto legislativo la cui efficacia è sospesa fino al 31 luglio 2007, non indispensabili per conseguire il risultato. È ovvio che tali norme, se accolta la proposta di stralcio, confluiranno - spero in un autonomo disegno di legge di cui il Governo si impegna a sollecitare la trattazione fin dalla ripresa autunnale dei lavori parlamentari. Si tratta di norme che possono richiedere uno sforzo di approfondimento da parte sia del Governo che del Parlamento, investendo aspetti importanti come l'assetto definitivo dell'organizzazione di tutti gli uffici giudiziari, ivi compresi quelli di procura ed i correlativi poteri del Consiglio superiore della magistratura e come la struttura stessa e l'organizzazione del Consiglio in relazione ai maggiori compiti connessi con la moltiplicazione dei momenti valutativi dei magistrati. In conclusione, onorevoli senatori, il provvedimento che stiamo esaminando non costituisce un'iniziativa volta a strutturare l'orditura ordinamentale a tutto vantaggio, come si è detto, della magistratura, tant'è vero che questi bagliori che ho richiamato annunciano uno sciopero che spero possa essere rimesso in maniera tale da consentire la serenità da parte del Parlamento, pur essendo evidentemente il Parlamento in grado di comporre debitamente questa annosa vertenza che da anni pone a disputa poteri dello Stato. Queste prese di posizione dimostrano che si tratta di un testo in cui sono compresenti le ragioni di tutte le componenti della società (ma la prima componente della società è quella che si chiama cittadino, persona); ragioni che non possono non essere tenute nella debita considerazione quando si operano modifiche destinate ad incidere su una parte fondamentale dell'organizzazione dello Stato e sono destinate ad incidere, direttamente o indirettamente, su diritti fondamentali dei cittadini, quello di essere giudicati da un giudice che sia autonomo, indipendente, imparziale e professionalmente adeguato. La conferma di ciò si ha solo si considera che i testi Castelli sono stati in parte conservati laddove le relative scelte di fondo erano ritenute corrette, talvolta rafforzandone la portata, come per l'accesso in magistratura e per il controllo costante sulla professionalità dei magistrati. Le modifiche più rilevanti sono state operate su aspetti della riforma che apparivano ai limiti della costituzionalità perché incidenti sull'autonomia e sull'indipendenza dell'ordine giudiziario; altre, le più numerose, attengono a profili di impraticabilità delle norme o sono dirette ad evitare effetti di ricaduta assolutamente negativi per lo stesso governo del corpo giudiziario, suscettibili di mettere in crisi - come ho detto all'inizio - la stessa attività del Consiglio superiore della magistratura. Mi auguro in conclusione, onorevoli senatori, che la discussione consenta lo scioglimento dei nodi politici che ci sono e che hanno fin qui caratterizzato l'*iter* parlamentare del provvedimento, al fine di consentirne un sereno esame e giungere finalmente alla sua approvazione. Ciò consentirebbe - credo - di chiudere definitivamente la stagione della contrapposizione in una materia vitale, quale quella della giustizia, e di garantire un quadro di riferimento stabile e condiviso per tutti gli operatori della giustizia, nel quale programmare e realizzare quei progetti essenziali per garantire al Paese una giurisdizione moderna, celere ed efficace. Le recenti sollecitazioni del Capo dello Stato erano del resto dirette proprio, da un lato, a ricordare l'urgenza di giungere ad una definizione della questione, ma anche, al tempo stesso, ad indicare l'esigenza di una soluzione il più possibile condivisa e stabile, dichiarando finalmente concluso il tempo delle ostilità tra poteri dello Stato. In questa linea mi sono sempre mosso secondo le mie ragioni, ma comprendendo quelle degli altri. Spero che queste ragioni (le nostre, quelle della magistratura e dell'avvocatura) siano comprese in questo provvedimento,

nell'amministrazione della giustizia italiana. Credo, onorevoli senatori, che quando avremo definito l'assetto dell'ordinamento, dovremo preoccuparci di evitare le lentezze, le lunghe procedure che non fanno dell'Italia quel grande Paese che è, rispetto al quale ognuno deve dare il proprio contributo autorevole dalla propria postazione di natura parlamentare e politica.

nel brusìo cacofonico dell'Aula; quindi, mi scuso se dirò qualcosa d'impreciso sulle dichiarazioni sia del relatore che del Ministro, ma ho inteso qualche sprazzo che mi ha colpito. Stavo anche riflettendo sul fatto che unanimemente si dice di questi tempi che la politica è debole. Mi sembra che proprio l'atteggiamento dell'Assemblea in questo momento abbia dimostrato, al di là di ogni dubbio, come la politica sia debole perché oggi noi perdiamo un ulteriore pezzo di sovranità - sto parlando del Parlamento determinando, almeno secondo la mia visione, un forte *vulnus* ai princìpi di Montesquieu nella più assoluta indifferenza dell'Assemblea. La politica dimostra quindi evidentemente una debolezza e una incapacità di capire quali sono i provvedimenti chiave per i quali il Parlamento abdica ai suoi poteri. Dall'andamento della discussione che si dipanerà in questi giorni potremo dimostrare questo nostro assunto.

una sorta di commedia, come cercherò di spiegare. Intanto mi ha colpito una frase del relatore. Ricordo che nella scorsa legislatura l'allora opposizione adduceva, come argomento per dimostrare che la nostra legge fosse sbagliata, che veniva attaccata da tutti;

caso, gli avvocati penalisti e i magistrati) fosse giusta. Ma vede, onorevole Di Lello, c'è una grossa differenza fra l'atteggiamento che assunse l'avvocatura e la magistratura per quanto riguarda la nostra legge rispetto alla vostra: sicuramente i penalisti fanno sciopero convintamente e rimpiangono il nostro testo; i magistrati, invece, fanno finta. Sono assolutamente convinto che la protesta dei magistrati sia finta, perché questa legge, come sa chiunque si intende di queste cose, non è nient'altro che il riassunto di due posizioni: le circolari del Consiglio superiore della

magistratura sono operazioni di alto valore istituzionale, trattandosi di un organo di rango costituzionale, ma nelle quali il Parlamento c'entra poco e nelle quali esso ha avuto un luogo meramente subalterno. Certo, anche questa è una scelta che l'Unione fa;

ci si arrende la guerra cessa, scoppia la pace, è normale. Lei, signor Ministro, si è arreso ancor prima di svolgere le sue funzioni. Ricordo che uno dei suoi primi atti è stato quello di recarsi, lei stesso, fatto assolutamente innovativo nella storia della Repubblica,

Chissà cosa diranno tutti i nostri partigiani che sono morti per la libertà: bastava che si arrendessero e non sarebbero morti, bastava che nessuno facesse resistenza e non ci sarebbero stati i lutti che ci sono stati. Bene, noi non condividiamo questo modo di pensare. Siamo del parere che, se una battaglia è ritenuta giusta, vale la pena di farla; è quella che abbiamo fatto nella scorsa legislatura, pagando anche dei prezzi personali, ed è quella che continueremo a fare in quest'Aula con i mezzi che il Regolamento e la democrazia ci consentono. Poi, evidentemente, prevarrà la forza e la logica dei numeri, anche perché, ripeto, credo - e del resto in qualche modo è inevitabile i colleghi che oggi seguono distrattamente o non seguono i nostri lavori, non riescono a rendersi conto di quanto grave sia la partita che si sta giocando in questo momento. La partita politica ed istituzionale è una sola

Visto che finiamo 1 a 1 chissà mai che i tempi supplementari, che si giocheranno nella prossima legislatura, non ci diano invece ulteriormente ragione. Per tali ragioni, invito i senatori, che peraltro giustamente hanno seguito distrattamente anche me

nel caso in cui il Parlamento, nel ramo del Senato, si risolva a votare un testo come quello proposto all'Aula dalla Commissione giustizia, dopo un esame, peraltro, assai approfondito e assai denso di proposizione e contrapposizione degli opposti argomenti su ogni singolo punto. Di fronte a

nel corso della XIV legislatura, quella riforma dell'ordinamento giudiziario che oggi è oggetto di controriforma. E vado con la memoria agli scioperi, in quella occasione indetti dall'Associazione nazionale magistrati. non riguardavano, signor Presidente, soltanto la riforma dell'ordinamento giudiziario ma qualunque batter di ciglia dell'allora maggioranza di centro-destra in materia di giustizia. Ricordo perfettamente le proteste, vivacissime e fortissime, dell'Associazione nazionale magistrati all'atto dell'introduzione del rito cosiddetto societario per regolare importanti e decisive per la nostra economia e per il nostro sviluppo economico. Ricordo le proteste vivacissime dell' Associazione nazionale magistrati al momento

la maggior parte delle quali sono oggi, tranquillamente ed efficacemente, in vigore. Alcune di queste proposte, invece, saranno state anche meritevoli di miglioramenti e correzioni, ma non meritavano certo che si urlasse allo scandalo.

di quelle prese di posizioni, meramente finalizzate a creare una contrapposizione solamente e strutturalmente politica nei confronti della maggioranza e del relativo Governo.

La conclusione, a ben pensare e a condizione di ben pensare, non può che essere questa. Il ragionamento non sarebbe completo se non fosse importata, nel perimetro dallo stesso disegnato, anche la malignità insinuata dal presidente Castelli secondo

argomento e possibilità di difesa a chi essa magistratura ha difeso. Ciò avviene attraverso un provvedimento che è la

Parlamento discusse della riforma dell'ordinamento giudiziario, ciò avvenne in varie successioni e per un tempo complessivo di tre anni e otto mesi. L'allora opposizione, oggi maggioranza, gridò

contingentati, non da lei, signor Presidente, ma dalla realtà dei fatti. La Commissione ha operato con la massima laboriosità possibile, ma ha avuto a disposizione un tempo complessivo di circa due mesi per esaminare un provvedimento per il

rispetto all'accordo politico che era stato disegnato nello scorso ottobre, quando il Governo ebbe la luce verde del Parlamento per potersi avviare verso un'operazione di controriforma (ne eravamo consapevoli allora e lo siamo ora), di quella parte dell'ordinamento giudiziario della riforma Castelli che non era in vigore. A noi sembra che questo tempo non sia

passaggi decisivi che oggi segnano un autentico ritorno al passato mi sembra obbligato e doveroso.

Ho chiesto di parlare su questo argomento perché, delle due argomentazioni fondamentali che sono contenute nella proposta del senatore Castelli, la prima ha forse soltanto un sapore, come suol dirsi, politico di reazione a discorsi che non abbiamo dimenticato, quando nella precedente legislatura si portava avanti - e si voleva arrivare fino in fondo

cioè una sorta di critica ad una legge, non per il suo contenuto, ma per il fatto che non risolveva tutti i problemi della giustizia. La risposta era che questa legge non era certo destinata a risolvere i problemi dei tempi della giustizia.

i pericoli per l'autonomia e l'indipendenza della magistratura (ma io ho voluto usare espressamente il termine giudice per le ragioni che dirò subito dopo); ragioni che dirò subito dopo); tale ritornello è ormai talmente ripetuto da avere creato una sorta di convincimento nell'opinione pubblica, invece è esattamente l'opposto.

che siedono ai banchi - oggi, della maggioranza - e che per anni si sono ripetutamente dichiarati gelosi custodi dell'indipendenza della magistratura e dei giudici

Invece, vi dico - anche per l'esperienza che ho potuto avere nella mia vita, proprio mentre sedevo nei banchi del Consiglio superiore della magistratura - che è esattamente il contrario.

avere il diritto di sovrapporsi al giudice che esercita attività giurisdizionale attraverso forme di monitoraggio, controllo e approvazione o non approvazione delle linee giurisdizionali seguite dai giudici. Questi, infatti, sono soggetti soltanto alla legge, perché tale è lo spirito della nostra Costituzione ed il valore fondamentale dell'indipendenza dei magistrati

sospensione e del suo ritorno in Commissione. Mi auguro, così, che vi sia un ripensamento che permetta di non far passare un provvedimento nel quale si stabilisce che, a partire da quando entrerà in vigore, chi va a fare il presidente di sezione di tribunale o il presidente di sezione di corte d'appello debba render conto delle proprie sentenze al Consiglio superiore della magistratura (cioè ad un organo che viene eletto

una rivendicazione dell'Associazione nazionale magistrati, pure molto sentita da tutta la magistratura italiana, ma che si tratta di cosa completamente diversa. Una cosa è una conferma condizionata all'approvazione di un organo estraneo, nel momento della fase del controllo dell'attività giurisdizionale, quando si esercita la funzione la funzione di giudice; una cosa è il controllo che si esprime non attraverso la conferma, ma attraverso la rotazione delle energie fresche, necessarie per evitare anche le cristallizzazioni di potere che

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: che all'articolo 3, comma 11, capoverso 17-*ter*, comma 1, vengano soppresse le parole da: "ovvero" fino alla fine del periodo; - che dopo il comma 29 dell'articolo 6 sia inserito il seguente; «29-*bis*. Le spese connesse alle disposizioni di cui ai commi 28 e 29 devono essere attuate nei limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura»; - che vengano soppressi i commi 33 e 34 dell'articolo 6; - che al comma 5, capoverso *o)*, dell'articolo 7, le parole: «ai commi 4 e 6», siano sostituite dalle altre: «al comma 6»; - che al comma 8 dell'articolo 8 siano soppresse le parole; «dell'articolo 4, commi 1 e 10»; - che all'articolo 9 venga introdotta una condizione volta a prevedere che dall'esercizio della delega non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Esprime, inoltre, parere contrario sul comma 35 dell'articolo 6. Esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 4, esprime poi parere non ostativo sulle proposte 3.107 e 3.110 a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, venga prevista una clausola volta ad escludere la corresponsione di compensi per la partecipazione al Comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura. Esprime altresì parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulle proposte 2.126, 2.128, 2.149, 2.150, 2.153 e 4.201. Esprime, infine, parere non ostativo sui restanti emendamenti».

è sicuramente l'articolo meno controverso di tutti quelli presenti nel disegno di legge Mastella, ma abbiamo ugualmente presentare alcuni emendamenti che sostanzialmente ricostituirebbero, se approvati, l'impianto originario della legge, che - ripeto - non è molto distante da quello attuale. Infatti, sulla questione dell'accesso alla magistratura sia l'attuale maggioranza che l'opposizione si sono trovate d'accordo sulla necessità di garantire un accesso cosiddetto di secondo livello. Ciò perché, evidentemente, si è riconosciuto il fatto che mettere nelle mani di ragazzi assolutamente preparati volenterosi, capaci, ma di poca esperienza una funzione così delicata come quella del magistrato

di altre esperienze di natura lavorativa, per trovarci di fronte a magistrati più preparati e più capaci di affrontare i loro delicati compiti. Ma allora perché proporre degli emendamenti e non lasciare il testo così come è, atteso che i cambiamenti, per così dire, non sono stati molti? Sostanzialmente per una questione: vorrei attirare l'attenzione dei colleghi su una questione che credo sia dirimente sotto questo punto di vista. Negli

durante l'esame di Stato vi fossero delle sedi in cui venivano tutti promossi - mi riferisco soprattutto ad alcune sedi del Sud - e altre sedi - soprattutto le sedi del Nord - in cui venivano sostanzialmente tutti bocciati. Giusto per capirci, a Catanzaro vi erano percentuali di promossi del 90 per cento, a Milano vi erano percentuali di bocciati dell'85 per cento. È chiaro che non può essere una questione di natura fisiologica, è chiaro che dal punto di vista statistico una situazione di questo genere non poteva essere realistica, però si creava un *vulnus* di natura costituzionale, cioè di ineguaglianza dei cittadini rispetto alle istituzioni. Chi nasceva al Nord evidentemente non era in grado di esercitare la funzione di avvocato, rispetto ad altri che invece avevano studiato in altre Regioni italiane. Questa distorsione ne ha creata un'altra di natura ancor più grave, il cosiddetto turismo forense: i ragazzi del Nord, vista l'impossibilità di passare gli esami a Milano, non facevano altro che iscriversi durante il tirocinio presso studi di Catanzaro e in questo modo assumevano il diritto di poter sostenere l'esame di accesso all'avvocatura a Catanzaro, superavano l'esame e potevano iniziare felicemente la carriera, creando però un *vulnus*. Addirittura in quella sede si era creata una vera e propria industria, che attraverso pacchetti ben definiti, garantiva il tirocinio e la promozione.

agli esempi che ha citato aggiungo anche l'intervento che abbiamo posto in essere - che tra l'altro doveva essere provvisorio, poi naturalmente come tutte le questioni provvisorie è diventato definitivo, di questo non si parla più credo giustamente credo giustamente - correggendo questa stortura. Oggi tutti i ragazzi italiani, tutti i giovani laureati in legge, hanno le stesse opportunità, gli stessi diritti, le stesse probabilità di accedere alla professione forense.

cento degli idonei è risultato appartenente alla città di Napoli. I napoletani sono certamente bravi, ma credo che anche tutti gli altri italiani siano bravi. È chiaro che dal punto di vista statistico è un dato che ci deve far pensare, è un dato che ci deve preoccupare; magari poi andando ad indagare non vi è nulla di distorto, però, insomma, è sicuramente un punto sul quale porre l'attenzione.

infatti possibile accedere direttamente alla carriera nel caso si sia laureati in facoltà evidentemente legate alla giurisprudenza e si sia sostenuto il dottorato di ricerca. Cosa c'entra questo con il discorso che sto facendo? C'entra, perché in questo Paese, uno strano Paese, che è centralista dal punto di vista nominale e ancora più ferocemente centralista dal punto di vista fiscale, in realtà, è non soltanto federalista, ma addirittura anarchico per quanto riguarda altre istituzioni, come le università. È noto che vi sono università in cui è difficilissimo

Questa fattispecie prevista oggi nel testo rischierà di ricreare tante "Catanzaro", questa volta non più per l'accesso all'avvocatura ma alla magistratura, perché ci saranno sicuramente università di serie B che per attirare studenti lascheranno ancora di più le maglie della loro severità, già in alcuni casi molto labile. Francamente non riesco a capire perché non si sia corretto questo aspetto in Commissione, che è evidente che non è né di destra né di sinistra;

che intervengono tutti su una questione che è stata oggetto di diffusa discussione nel corso dei lavori della Commissione e che continua, a mio modo di vedere, a non trovare una soddisfacente risposta. Si tratta della questione "almeno di norma", con riferimento al momento in cui devono essere banditi i concorsi per l'accesso in magistratura. Riepilogo la questione per migliore comprensione mia e dei colleghi. Nel testo originario proposto dal Governo si diceva che i concorsi sono banditi almeno una volta all'anno. Dietro a all'espressione

i concorsi tutte le volte che è necessario. Chi ha presentato tale emendamento si chiede perché ingessare il Ministro della giustizia vincolandolo a un numero preciso.

Pur riservando parole di apprezzamento all'una e all'altra soluzione, trovo che tuttavia la soluzione adottata non sia né convincente né adeguata, per una questione che - badate bene - è delicatissima. il numero di nuovi magistrati che vengono introdotti nel sistema non è un numero di soggetti semplicemente destinato alla funzione giudiziaria. Occorre che su questo facciamo un esercizio di realismo e di trasparenza molto chiaro. Fino a quando l'attuale sistema e l'attuale assetto saranno quelli di un Consiglio superiore della magistratura che è la rappresentazione dell'Associazione nazionale magistrati, o meglio

in un momento piuttosto che nell'altro, in una scadenza elettorale piuttosto che in un'altra, in una congiuntura piuttosto che in un'altra, è destinata a drogare il sistema. Ciò non è opportuno e non è utile, perché quanto vi sto rappresentando, signor Presidente, non è uno degli aspetti più virtuosi del nostro sistema giudiziario. Di qui la necessità che quantomeno il momento dell'accesso in magistratura, che decorre necessariamente e fisiologicamente con il momento in cui è bandito il concorso, sia sottratto alla responsabilità di individuazione da parte del Ministro, me ne sarà grato. Ciò vorrà dire liberarsi di una responsabilità di rilievo e di un sospetto sempre possibile di rilievo, e deve essere a data fissa data fissa e legato a un evento che non possa essere modificato dai fatti. L'unico evento che mi è venuto in mente è quello del raggiungimento di un determinato *quorum* dei posti che si rendono vacanti (o che sono vacanti) secondo la prospettazione voluta dal Governo. Ho quindi presentato vari emendamenti, che tra l'altro sono variabili solamente nel numero: se sarà accolto il sistema, saranno uno preclusivo di tutti gli altri, se il sistema non sarà accolto, ritirerò volentieri quelli restanti. Ho voluto lasciare al sottosegretario Scotti,

Presidente, il tema è quello che è stato trattato poc'anzi dal senatore Caruso; rilevo l'ineffabilità della proposta legislativa nel momento in cui la legge non è in grado di stabilire quante volte si debba fare un concorso, se si debba fare una volta l'anno o due volte l'anno, oppure ogni due anni: questo di norma è un termine troppo elastico per poter essere introdotto un disegno di legge che fisiologicamente deve essere rigoroso. Rassegno questo alla valutazione dell'Assemblea: si dica quante volte si debba fare un concorso, oppure si tenga conto di quei parametri che così opportunamente ha introdotto poc'anzi nel dibattito, illustrando i propri emendamenti, il senatore Caruso, ma non si può restare ancorati all'ineffabile, a questa approssimazione. Una legge ha il diritto di essere puntuale e rigorosa, e così non è.

propone di introdurre una normativa che regoli la cadenza delle prove. Nella legge viene indicato quali sono le prove, manca però un'indicazione del modo con cui si proporranno ai concorrenti.

siamo anche disponibili a indicarlo per legge preventivamente, al momento in cui viene bandito il concorso, oppure attraverso una preventiva indicazione della sequenza. Penso che comunque sia importante questo tipo di introduzione per non lasciare monca la disposizione ai fini dell'elencazione della sequenza.

nell'ambito della pubblica amministrazione, non si possano sommare più anzianità che sono state maturate in settori diversi della pubblica amministrazione. Se si è passati, attraverso la mobilità, dall'amministrazione dell'interno all'amministrazione della giustizia e si hanno i requisiti, sommando gli anni necessari, non si comprende perché non si possa partecipare poi al concorso e si debbano avere quegli anni solo ed esclusivamente in un unico ramo della pubblica amministrazione. Non riesco comprendere, se il requisito è quello della laurea, di una certa fascia dirigenziale

vorrei chiarire subito ai colleghi che gli emendamenti che ho presentato all'articolo 1 del testo sono di carattere strutturale. Tendono semplicemente a correggere quelli che a me sembrano degli errori nell'impianto formulato e non hanno, sotto questo profilo, alcuna rilevanza politica tale da suscitare le ire dei magistrati, i quali - apro e chiudo una parentesi, signor Ministro - hanno testé proclamato uno sciopero per il 20 luglio; la qualcosa, devo dire la verità, ci appare singolare, nel senso che, come vede (gli era stato già detto in altre occasioni), lei può fare tutti gli sforzi che vuole, ma come si distanzia solo un millimetro dalle posizioni dei magistrati, ahimè, anche lei, da loro così ben voluto, non può essere di ostacolo alla proclamazione dello sciopero. sciopero. Gli emendamenti da me presentati hanno un carattere non politico, ma semplicemente strutturale. Li tratterò in maniera più specifica nell'ambito della dichiarazione di voto; certo è, però, che davvero non si comprende, ad esempio, come all'interno delle categorie che vengono individuate come idonee al concorso in magistratura vi siano rilevanti disparità di trattamento. Ad esempio, non si comprende la ragione per la quale chi ha vinto un concorso nello Stato in area dirigenziale e presta servizio per quattro anni, invece che i cinque previsti nel testo, non può fare il concorso in magistratura, mentre lo può fare un non meglio specificato personale docente in materie giuridiche, indipendentemente dall'anzianità di servizio. Ancora, Presidente, alcuni emendamenti riguardano il logistico del concorso in magistratura; in particolare, la previsione che il concorso in magistratura, per ragioni evidenti di praticità, possa svolgersi in più sedi. Questa previsione ci preoccupa, anche perché l'esperienza pregressa concernente gli esami per procuratore o per avvocato ci ha convinto che la differenza delle sedi è particolarmente rilevante in quanto, in genere, molto diverso è il tipo di sorveglianza che in quelle sedi viene effettuata. E, d'altra parte, Presidente, non potendoci pensare, ancorandomi all'esperienza che tutti quelli che che facevano l'esame di procuratore in una determinata città erano dei geni, a differenza di altri che facendolo in un'altra tanto geni non erano, perché le statistiche di bocciatura e di promozione parlavano da sole, devo dire che, evidentemente, la differenza dei risultati non era dovuta tanto alla capacità giuridica dei soggetti, ma alla differenza della sorveglianza. sorveglianza. A me pare che immaginare più sedi significa anche immaginare diversità di sorveglianza. Una cosa voglio dire al relatore, al Ministro e ai colleghi, per quello che vale. Avendo immaginato questo concorso come un concorso di secondo grado, non ci sarà più quella folla scatenata che c'è stata fino adesso di candidati al concorso in magistratura. È chiaro, infatti, che fino a quando il concorso in magistratura era accessibile da chi aveva solo il diploma di laurea, il numero dei candidati era sicuramente diverso

che, in caso di parità, prevalga il voto del presidente o del magistrato più anziano, teoricamente si potrebbe consentire una valutazione non a tre, ma a due. Sottosegretario Scotti, come ella sa molto meglio di me, che questi sottocomitati vengono considerati dalla giustizia amministrativa dei collegi perfetti; sembra pertanto singolare che nella norma si inserisca una disposizione in contrasto con la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato.

solo per segnalare che un vostro gentilissimo ed efficiente funzionario mi ha fatto notare che, per mantenere in vita

Desidero resti agli atti che si tratta di un cambiamento solo di natura tecnica perché sono convinto che il testo precedente fosse, almeno da un punto di vista sostanziale, sicuramente migliore perché francamente queste variazioni di natura semantica non mi hanno mai convinto; però, il Governo e la maggioranza hanno voluto introdurre anche una novità di questa natura di cui prendo atto.

*(AN)*. Presidente, intervengo per dichiarare il voto, che sarà ovviamente a favore, del Gruppo di Alleanza Nazionale sull'emendamento 1.200. Se lo stesso fosse accolto, va da sé che saranno preclusi tutti gli altri. Se lo stesso non sarà accolto, in coerenza con quello che ho dichiarato prima e solo per questa ragione annuncio il ritiro degli emendamenti che intervengono sullo stesso argomento, togliendole così il disturbo di fare questo minimo cangurino che lei ha annunciato. annunciato. Il silenzio del Ministro, il silenzio del Sottosegretario e il silenzio del relatore nel tentare un abbozzo di argomentazione al parere contrario su questo emendamento e su questa proposta,

sulla fondatezza di quel sospetto evocato nel corso dell'illustrazione della questione del non passaggio all'esame degli articoli da parte del presidente Castelli e da me ricordato. Questo non è il parere del Ministro; questo non è il parere del Sottosegretario; questo non è il parere del relatore; questo è il parere di chi ha paura che venga introdotto un parametro di trasparenza in una questione delicata, qual è quella dell'accesso di nuove risorse alla magistratura. Questo è il parere più deteriore delle correnti dell'Associazione nazionale magistrati.

si potrà avere la possibilità che preventivamente si possano chiudere quei posti vacanti nel ruolo della magistratura che, ogni anno, registra assenze

ci sarà una cadenza annuale in grado di andare a copertura costante e continua dei posti che sono rimasti vacanti. Non si capisce perché

risultare vacanti successivamente poca importanza aveva. In realtà, qui si introduce un parametro obiettivo che consente un meccanismo automatico. Non vi è una necessità di prevedere e di verificare se dobbiamo fare un concorso per 300, 400, 500 posti o addirittura due concorsi nello stesso anno. Attraverso un meccanismo automatico, la magistratura sa che comunque ci sarà un ingresso in automatico di tot numero di magistrati ogni anno; si potranno regolare le vacanze e quindi si potrà avere la possibilità di evitare che quelle vacanze durino più del tempo necessario a causa del tirocinio che comunque ha la sua durata, a causa della necessità di coprire quei posti attraverso una previsione automatica. Francamente è incomprensibile. Anche questo forse risponde a logiche di potere che devono controllare persino quanti posti bisogna mettere a concorso. Siamo arrivati all'assurdo e oltre i limiti del comprensibile per il buon andamento della pubblica amministrazione.

già esposto dai colleghi Centaro e Caruso, dicendo che le condivido pienamente. Non si riesce a capire perché una norma così banale e di buon senso non viene recepita se non per evidenti ed inconfessabili retropensieri. Vi è però anche una questione di natura formale, sulla quale credo che la Presidenza dovrebbe porsi il problema e così tutti noi che dovremmo avere una dignità dei legislatori. Che senso ha dettare norme di questa natura? Scrivere che un concorso si tiene "con cadenza di norma annuale" significa non scrivere nulla.

sia una presa in giro per i cittadini che il legislatore possa scrivere una norma che sa *a priori* essere priva di qualsiasi significato. Vi sono emendamenti dichiarati privi di innovazione. Mi sembra che dovremmo porre questa problematica anche sui testi di legge: questa è una norma priva di qualsiasi innovazione.

Presidente, le chiedo scusa, ma non mi sono espresso in maniera sufficientemente chiara: sono ritirati - e sono gli unici che saranno ritirati - tutti gli emendamenti che affrontano il problema della trasparenza nel

Presidente, continuo a non comprendere le ragioni della contrarietà all'emendamento 1.101, considerato che comunque nel testo di legge un metodo di sequenza delle prove va indicato; che poi sia una sequenza preventivamente preordinata, indicata anche nel bando di concorso, oppure, come avviene oggi, una sequenza sorteggiata il giorno della prova, proprio per far sì che comunque i candidati non abbiano

con l'approfondimento, così recita il testo proposto, dei temi della concorrenza, della contraffazione e della tutela dei consumatori. Nel corso dell'intervento generale precedente, ho ricordato ai colleghi dell'Assemblea che quella che viene celebrata oggi è una cerimonia che secondo la nostra Costituzione doveva essere celebrata sessant'anni fa. Mi sembra che il gravissimo ritardo con il quale il Parlamento, dopo i batti e ribatti della riforma proposta dal ministro Castelli e votata

in precedenza. Queste materie non attengono soltanto alla problematica civile, ma anche a quella penale, in virtù del proliferare di una normativa sanzionatoria sempre più forte

evoluzione della preparazione della magistratura, ad una maggiore qualificazione, alla possibilità di rendersi conto dell'evoluzione dei tempi e, quindi, di sfornare magistrati veramente all'altezza del loro compito.

dal punto di vista del legislatore, dovrebbe restare in vigore per molti anni. Quindi, non possiamo

In questo caso, addirittura, non soltanto non ci preoccupiamo del futuro, ma ignoriamo anche il presente. Quante volte abbiamo detto in convegni, interviste, articoli, che la competitività di un Paese è legata alla sua capacità di costruire brevetti ed innovazioni, di innovare cioè i prodotti che pone sul mercato globalizzato? Quante volte ci siamo detti che esiste il problema della contraffazione? Oggi, infatti, Stati enormi come la Cina, che hanno una capacità produttiva

dichiara che c'è stata effettivamente una violazione in materia brevettuale o di diritto d'autore, di fatto emette la sentenza, perché è rarissimo il caso - e per

ancorati ai vecchi schematismi del diritto e non si è avuto il coraggio di introdurre una minima innovazione. Tutto ciò sta a dimostrazione di come non si stia varando una riforma nel senso della modernità,

La figura del consulente è importante, dà un contributo di modernità, di attualità, di rigore scientifico ai temi sottoposti alla sua valutazione. Pertanto, ritengo che questo studio, che fatalmente sarebbe effimero e superficiale, non possa sostituire la valutazione pregnante e rigorosa del consulente. Credo quindi che, sotto questo profilo, l'emendamento 1.207, con tutto il rispetto e la stima per chi lo ha steso, non meriti di essere considerato con particolare attenzione. Per tale ragione, voterò in dissenso

abbiamo di fronte tre prove scritte, pagate con 12 ventesimi per conseguire la sufficienza, il cui Poi, abbiamo dieci prove orali, pagate - chiedo ancora scusa per la rozzezza dell'espressione - con sei decimi: viene modificato il sistema di sufficienza, di sufficienza, che, in tutte le prove orali, si consegue con 60 centesimi: 60 + 36 fa 96. Resta la previsione contenuta nella lettera cioè un giudizio di sufficienza in quello che la disposizione recita essere un colloquio - quindi, certamente non una prova scritta - in una delle lingue straniere indicate dal candidato, che dovrebbe essere ragionevolmente pagato con sei decimi. Se così è, il totale a cui nel suo riconteggio avrebbe dovuto pervenire il valoroso relatore sarebbe stato 102 e non 108. Voterò a favore dell'emendamento 1.102 soltanto se il relatore

di fronte alla saggezza dei colleghi (di maggioranza, intendo dire), ma per il fatto che, siccome è stata appena votato una norma che stabilisce l'impossibilità di essere sufficienti all'esame, sarebbe assolutamente contraddittorio se il Senato volesse accettare l'idea di approfondire e controllare la capacità psico-attitudinale dei candidati.

voterò a favore di questo emendamento e raccomando ai colleghi del mio Gruppo di fare altrettanto, ma non posso che rassegnarmi al relativo esito. Presidente, Forza Italia voterà a favore dell'emendamento 1.208, che tanto scandalo ha suscitato nella magistratura italiana: vengono evocate dichiarazioni certamente travisate e modificate da un impianto mediatico (favorevole, come sempre, al centro-sinistra), ma, in realtà, ciò che si chiede è una valutazione complessiva di idoneità psicofisica di una persona che si approssima a svolgere una funzione di straordinaria delicatezza. Non si comprende perché chi deve accedere ad un'attività nell'ambito delle forze dell'ordine o dell'Esercito debba superare questo tipo di prove e non un magistrato. Mi si risponde che in realtà costoro avranno il maneggio della pistola, di un'arma che comunque può colpire, può danneggiare, può uccidere, e così il magistrato, attraverso la penna, maneggia la vita degli altri cittadini attraverso le ordinanze di custodia cautelare e può incidere sulla vita, sulla salute e sul patrimonio dei cittadini, con conseguenze spesso molto ma molto più devastanti di un colpo pistola. Ci dobbiamo allora intendere. Qui non si vuole

mentale; dunque, anche i magistrati possono preventivamente subire un esame che è in tutta evidenza assolutamente superficiale: nessuno andrà a fare

Torno a dire che non c'è alcuna voglia di penalizzare nessuno e d'altra parte in questo caso siamo nella fase preliminare di accesso al concorso. Dio solo sa quante volte il Consiglio superiore della magistratura è dovuto intervenire per sanare vere e proprie follie, come quelle di magistrati che facevano il tiro a segno con la pistola negli archivi sotterranei dei tribunali o di coloro che andavano in giro in mutande, coperti solo dalla toga. toga. Tutto questo dà conto di una situazione che capita in tutte le categorie: potrei fare un'elencazione particolarmente colorita e suggestiva in virtù delle esperienze svolte. Penso allora che sia comunque importante

Ritengo invece che dopo un periodo di attività in un contesto tutto particolare, qual è la magistratura, dove si può verificare una serie di condizionamenti, di esaltazioni, di rapporti atipici con la realtà, oltre che naturalmente di corretta interlocuzione con i problemi con i quali ci si deve confrontare,

attualmente sospeso completamente travisata dall'ordine della magistratura.

vittoria del concorso, persone che possono anche essere psicologicamente e psichicamente labili. Chiunque abbia avuto a che fare con l'attività del Ministero lo sa: purtroppo nascono

relativo alla capacità e alle grandi doti di equilibrio che un magistrato deve possedere e che in qualche modo sembra fossero messe in dubbio

che prima di estrinsecarsi in tutta la loro evidenza hanno avuto un periodo di incubazione in cui il magistrato in tribunale compie delle assolute stranezze. Potrei dilungarmi su esempi clamorosi da questo punto di vista. È evidente che, sia gli avvocati, sia i colleghi, sia soprattutto i cittadini che non conoscono questo quadro e vedono comunque il magistrato attivo negli uffici giudiziari, hanno un'immagine della magistratura che evidentemente va a disdoro della carriera stessa. Si era posto, quindi, questo filtro per evitare che costoro potessero esercitare le delicatissime funzioni di magistrato. Invece, tutto ciò è stato interpretato in maniera esattamente contraria; quindi, l'ANM, che ha scritto questo testo, come dimostra anche la parte ora in esame, ha preteso la cancellazione di quel passaggio, a mio parere, in maniera autolesionistica, perché in questo modo statuisce la possibilità di accesso alla magistratura anche per soggetti psicologicamente instabili. Nulla vieta, infatti, che un soggetto psicologicamente instabile sia intelligente e colto al punto di poter superare il concorso. ciò - ripeto - non potrà che riverberarsi in un *vulnus* per l'immagine stessa della magistratura, perché senza nessun filtro inevitabilmente questi casi si ripeteranno ripeteranno in futuro. Sono convinto che probabilmente anche in questo momento il ministro Mastella ha a che fare con qualche caso di questa natura, è statisticamente inevitabile, mentre si potrebbe evitare

Signor Presidente, sempre a causa dell'improvvida approvazione da parte del Senato dell'emendamento 1.102, è probabile che non vi sia un grande numero di partecipanti al concorso per l'accesso in magistratura i quali, pur essendo risultati idonei a fronte del superamento di tutte le prove scritte e orali, tuttavia non abbiano un punteggio sufficiente per poter entrare in graduatoria ed essere quindi nominati magistrati. Occorre dire che, paradossalmente, quell'errore prima compiuto dal relatore e confermato dal Senato ha l'effetto di ridurre il problema che tuttavia comunque esiste. esiste. Il testo proposto dal ministro Mastella contiene un'aria di cattiveria nei confronti di tutti coloro i quali, pur essendo risultati idonei nel concorso, concorso, non vedranno tenere nel minimo conto la loro idoneità nei concorsi successivi a cui essi dovessero partecipare, ancorché immediatamente prossimi a quello in cui, malgrado l'idoneità, non abbiano potuto conseguire l'auspicato risultato. Si è detto, con questa cultura del sospetto che un po' ha caratterizzato i lavori

a questo aspetto del problema: è mio costume pensare che coloro i quali si differenziano da altri per oggettive ragioni comunque devono veder corrispondere questa differenziazione anche ad un difforme trattamento. Questo all'emendamento 1.209 in discussione, che, per l'appunto, prevede che siano direttamente ammessi alla prova orale, saltando quindi l'alea della prova scritta, coloro i quali, idonei, non abbiamo raggiunto un punteggio sufficiente per poter essere nominati magistrati. Questo, come dicevo, non in termini assoluti, ma solo con riferimento ad uno dei due concorsi immediatamente precedenti a quello a cui il candidato intende nuovamente partecipare. Mi sembra una norma di equità sostanziale, di semplificazione dei rapporti tra lo Stato e gli aspiranti partecipi all'apparato dello Stato; mi sembra, fra l'altro, una di quelle norme che servono a ridurre significativamente il contenzioso che, come noi ben sappiamo, come sanno coloro che in particolare hanno avuto esperienze di Governo, caratterizza i concorsi per l'accesso in magistratura; ne sono stati oggetto sistematico nel passato i cosiddetti *quiz* che costituivano la prova di preselezione per il concorso, ne costituiranno in questo caso il presupposto i concorsi stessi.

mi è stato recapitato un testo che ha l'aspetto di un emendamento, anzi è anche numerato come tale (2.134), che però porta la firma di un senatore,

Gruppo di Forza Italia voterà a favore di questo emendamento che francamente mi meraviglia molto non venga accolto dal relatore e dal Governo, perché si verifica una vicenda strana: un soggetto riesce ad avere l'idoneità, e quindi quel punteggio minimo o più che minimo sufficiente a fargli superare il concorso, in quanto è stato già dichiarato idoneo, con una evenienza negativa derivante dalla circostanza che, ad esempio, per un concorso a 400 posti, ne vengano dichiarati idonei 450. Gli ultimi 50 in graduatoria come punteggio ottenuto, pur essendo stati dichiarati idonei in quanto hanno superato quel minimo necessario per poter essere dichiarati tali, rimangono assolutamente fuori. A volte si verificano evenienze positive e più fortunate, nel senso che non vengono neppure coperti tutti i posti messi a concorso; altre volte vi è un numero di idonei di gran lunga superiore. Mi chiedo: visto che costoro hanno comunque superato le prove a quel livello ritenuto sufficiente per essere dichiarati idonei e, quindi, per essere assunti in magistratura, perché devono rifare totalmente il concorso e non devono avere almeno l'agevolazione derivante dalla circostanza che possono accedere direttamente alle prove orali, quando, torno a dire, costoro hanno superato sia le prove scritte che le prove orali con un punteggio tale da farli riconoscere idonei e quindi con un'evenienza più favorevole, non farli rientrare nel novero dei magistrati da assumere? Questa chiusura assolutamente incomprensibile e punitiva nei confronti di persone che, comunque, hanno già dimostrato di essere all'altezza, sotto il profilo del punteggio, di accedere alla magistratura.

credo che sia il senatore Caruso che il senatore Centaro abbiano addotto delle argomentazioni di assoluto buon senso, che non sono nemmeno ascrivibili ad una visione visione sull'andamento della giurisdizione che possa essere di destra o di sinistra; semplicemente portano avanti un'argomentazione in difesa di quegli aspiranti che hanno superato l'esame e sono stati dichiarati idonei. Ho già fatto rilevare la circostanza del tutto anomala che a rappresentare il Governo oggi c'è il Ministro, ma credo più che altro in funzione di senatore, visto che il suo voto è fondamentale, e quindi continuo - non me ne voglia il Ministro a pensare che sulla materia il Governo è rappresentato dal sottosegretario Scotti. Sottosegretario Scotti, lei (l'ho già rilevato più volte e la mia rilevazione prescinde ovviamente dalla sua persona: è un'annotazione di natura politico-istituzionale) non è neanche senatore, è stato paracadutato in questa sede dai magistrati da magistrato; lei è un magistrato a tutti gli effetti ed è stato messo qui per sorvegliare che i senatori non tralignino e che, quindi, portino avanti in maniera assolutamente

per rispetto all'Aula, di dichiarare perché il Governo si dichiara contrario a questi emendamenti. Accontentatevi della grande vittoria che avete imposto a quest'Aula imponendo i vostri testi, ma almeno non umiliateci; fateci capire perché certe proposte di assoluto buonsenso vengono respinte.

sull'ordine dei lavori: prima erroneamente ho votato in maniera diversa da quanto ho dichiarato, per un errore materiale, ma il mio voto nella votazione precedente sarebbe da registrare come voto di astensione; adesso starò più attento. Per quanto riguarda l'emendamento 1.209, sono in dissenso da quanto espresso dal mio Gruppo attraverso l'intervento del presidente Castelli, che peraltro ha spiegato esaustivamente il contenuto dell'emendamento stesso, perché come ritengo che un controllo psico-attitudinale sia non solo indispensabile, ma debba anche essere ripetuto periodicamente nel tempo, così credo che la questione dei concorsi andrebbe integralmente rivista, nel senso che abbiamo registrato in passato, ma anche recentemente, situazioni che hanno dimostrato come l'attuale modalità di selezione dei magistrati sia assolutamente inadeguata. Alla fine, con un semplice concorso per titoli e per prove, per prove, persone da poco laureate, con un'esperienza lavorativa e, diciamo pure, di vita sociale nel suo complesso estremamente limitata, si trovano catapultate in situazioni estremamente delicate e sono nella condizione di poter poter decidere letteralmente della vita delle persone, degli altri cittadini con risultati che spesso lasciano a desiderare. Da Da parte dell'Associazione nazionale magistrati, quindi, non ci dovrebbe essere un atteggiamento come quello che stiamo vedendo in quest'Aula, di imposizione di alcuni punti di vista, fino ad arrivare a scrivere, se non le leggi nel loro complesso, comunque parti importanti delle stesse, come interi

Presidente, sembra una grossa contraddizione procedere in questo modo con i lavori.

un voto di laurea non inferiore a 107 centodecimi per poter vantare i requisiti per iscriversi al concorso in magistratura.

finito un percorso universitario, riescono ad ottenere il dottorato di ricerca. Si tratta di studenti che lavorano sui testi, approfondiscono materie giuridiche, aiutano

l'associazione spontanea nata tra i dottori di ricerca (i famosi *PhD*, riconosciuti in tutta Europa e in tutto il mondo) stia facendo anche pressione verso

Ma andiamo avanti. Perché non si possono ammettere o con quale motivazione si può escludere chi già ha ottenuto l'abilitazione alla professione forense che potrebbe, pertanto, esercitare la professione di avvocato,

conferisce un'abilitazione? Perché non poteva essere inserito questo emendamento come un emendamento intelligente? Arriviamo all'ultima delle tre questioni sollevate da questo emendamento:

è derivante non da colpa propria, ma dal non poter permettersi di avere la scienza infusa e di conoscere l'universo mondo, tutte le discipline e tutte le materie che vengono loro sottoposte e soprattutto una: l'imponente macchina

la grande conoscenza del diritto amministrativo e dell'operare della pubblica amministrazione veniva considerato sufficiente a conferire una qualifica di arbitro, seppur in quel caso onorario. onorario. Guardate, è già stato detto che alla fine i giudici non decideranno più nulla, saranno costretti, ogni qual volta si troveranno di fronte a casi determinati e a materie particolarmente ostiche, tra le quali la conoscenza della pubblica amministrazione, a nominare

aspetti sostanzialmente tecnici a personale non appartenente alla magistratura per l'impossibilità di conoscere da parte del magistrato. C'è addirittura una corrente di pensiero che va contro la gradualità della carriera dei magistrati, perché un giovane

popolare da suggerire che l'ingresso non sia come giudice monocratico di primo grado, ma addirittura come una parificata posizione

sottosegretario Scotti, sottolineo che quello che si propone con questi emendamenti, che tendono a modificare in senso ragionevole,

affermazione mi ha un pochino sorpreso. Non so se il suo sia un *pluralis modestiae* o un *pluralis maiestatis* perché, per quanto mi riguarda, non credo si riferisca a nessun organismo di natura collegiale perché non ricordo - sono stato a quasi tutte le Conferenze dei Capigruppo - che si sia raggiunto un *gentlemen agreement* di questa natura. Il fatto che il *fair play* dell'opposizione

attenersi al Regolamento, atteso che una norma di questo genere, a cui lei si è richiamato, può essere viva solo in caso di accordo anche di chi la subisce. Se però il senatore Galli o qualsiasi altro mio collega - parlo ovviamente per il mio Gruppo

la convenzione vissuta in quest'Aula da quasi l'inizio della legislatura è vero, come lei ha detto, che non abbiamo mai fatto riferimento a ciò nella Conferenza dei Capigruppo. Ma è altrettanto vero che da lungo tempo in quest'Aula, quindi con il silenzio-assenso anche del Gruppo che lei presiede, abbiamo adottato questa prassi, questa prassi, della quale io in questo momento, ma anche altri Vice presidenti si sono avvalsi, utilizzando, tra l'altro, una norma regolamentare, prevista esattamente dall'articolo 84, che conferisce alla Presidenza del Senato la facoltà di armonizzare i lavori dell'Assemblea in relazione ai tempi più o meno elastici che ci siamo dati e che abbiamo convenuto per quanto riguarda il percorso d'Aula di questo provvedimento. senatore Castelli, che questa facoltà è propria della Presidenza, che la utilizzerà nel modo più elastico possibile per venire incontro alle esigenze dei Gruppi, anche di quei colleghi ovviamente che si pronunciano in dissenso, preservando però l'obiettivo che nella Conferenza dei Capigruppo ci siamo dati di approvare il provvedimento entro la settimana, anche andando ad un'eventuale seduta sabato mattina.

Presidente, credo che la consuetudine che si è creata all'interno di quest'Aula non sia voluta, ma legata al fatto che la stragrande maggioranza dei provvedimenti che qui abbiamo esaminato o avevano una scadenza

No, senatore Calderoli, perché questa mattina nella Conferenza dei Capigruppo, in realtà, con il consenso di tutti, abbiamo previsto un'armonizzazione complessiva dei tempi per l'approvazione di questo provvedimento nella settimana in il Presidente una notevole opposizione da una parte dei rappresentanti dell'opposizione e anche delle dichiarazioni in dissenso, si debba pervenire ad un equilibrio tra le possibilità e le facoltà dei Gruppi parlamentari e dei singoli senatori e senatrici di intervenire anche in dissenso su tutto il provvedimento. Quindi, un minimo di armonizzazione, prevista già dalla fase iniziale, mi sembra necessaria. Presidente, cedo alla violenza, però, se il Presidente del Senato ha detto che avremmo valutato domani eventuali modalità di armonizzazione, (alle quali ci siamo preventivamente dichiarati contrari),

senatore Calderoli, a parte il fatto che tutti i senatori hanno il diritto di parlare eventualmente anche in dissenso rispetto al loro Gruppo, io questo diritto lo devo comunque preservare verifica in sede di Conferenza dei Capigruppo per domani mattina sull'andamento dei nostri lavori era dovuta non alla questione sollevata dal collega Galli e dal collega Castelli, ma ad un'eventuale nuova iniziativa da parte del Governo,

Presidente, questo emendamento si propone di consentire la somma degli anni trascorsi nella pubblica amministrazione a coloro che vogliono accedere al concorso. È prevista separata per coloro che sono laureati in legge, che abbiano un certo livello di qualifica dirigenziale e abbiano conseguito un certo numero di anni di servizio nelle funzioni svolte all'interno della pubblica amministrazione: mi chiedo per quale motivo non si possano sommare

costoro debbano aspettare di maturare i cinque anni, per esempio presso l'Amministrazione della giustizia o altrove per poter disporre di questa via privilegiata al concorso. Non si sta chiedendo nulla di particolare o accessi privilegiati, ma semplicemente di conteggiare gli anni trascorsi in rami diversi della pubblica amministrazione ai fini di quella sommatoria finale.

se il superamento di una prova quale il dottorato di ricerca non esistesse; come se il superamento di un esame di abilitazione alla carriera forense non contasse assolutamente niente.

alla carriera magistratuale studenti che provenivano da università dove tale valutazione era tenuta con un margine di valutazione migliore. Il Ministro però ha dovuto accettare che la Commissione eliminasse l'inserimento

si possano fare ragionamenti di buon senso in tutte le direzioni. Ricordo però che in un Parlamento dove si approvano le leggi io rappresento una parte del Paese che evidentemente è in dissenso con chi rappresenta coloro i quali hanno dato il voto a chi governa;

nell'immissione in ruolo dei magistrati, perché chiaramente certe situazioni che si vengono a creare dipendono anche dal tipo di preparazione che consente a queste persone di diventare magistrati.

uno dei punti dell'Ulivo - qualificante - era rendere veramente qualcosa in più rispetto al centro‑destra. E allora, vedo uno stato di sofferenza: un contatto tra le manifestazioni

È per questo che il mio voto di astensione arriva in un momento - proprio così - di sofferenza, avendo inoltre simpatia per il ministro Mastella, perché occupa - non dico militarmente, ma grazie al suo grosso peso - il posto del presidente Prodi. questa simpatia, dall'inizio della discussione, mi porta con umiltà, ma anche con molta determinazione, a rinnovare il mio voto di astensione, che è ‑ lo ribadisco ‑ un voto di simpatia. Purtroppo, devo dire che forse il dibattito non ha appassionato molto quest'Aula, perché, alla fine, invece della riforma mi sembra si sia partorito un topolino,

questo passaggio fondamentale in cui si determinano i soggetti ammessi all'esame. Dobbiamo riflettere attentamente prima di prendere una decisione che vada nel senso auspicato dai proponenti dell'emendamento,

una platea più ampia e vasta di partecipare a questi esami. Credo sia davvero assolutamente necessario che l'Aula rifletta su questo aspetto. Io porto la mia personale

Il solerte dottor Castiglia, come suo dovere, le ha fatto notare quell'articolo del Regolamento - peraltro ben noto a tutti - in base al quale il Presidente di turno è autorizzato

chiaro, in modo che il mio pensiero le giunga inequivocabilmente: lei non ha diritto a coartare il Regolamento. È del tutto evidente che la sua facoltà di interrompere i colleghi vale se siamo d'accordo, ma non vale se non siamo d'accordo: su questo non vi è il minimo dubbio.

Anch'io, signor Presidente, voterò in dissenso dal mio Gruppo e colgo l'occasione, però, per

tanto che ne porto ancora le conseguenze, per così dire. Appena diventato consigliere comunale per il mio movimento - sono stato il primo, lo voglio ricordare, correva l'anno 1985- dopo il primo Consiglio comunale, sono stato chiamato da un magistrato di Varese a rendere conto delle dichiarazioni fatte in Consiglio comunale. Mi ero Mi ero limitato a dire che volevo che il Consiglio comunale si dotasse un nuovo Regolamento per l'assegnazione delle case popolari,

manifestazione di idee illegali, aveva pensato bene di iscrivermi nel registro degli indagati. Sulla base di queste situazioni che

Devo anche ricordare che il mio segretario federale, onorevole Bossi, sta pagando ancora oggi, con una ritenuta sulla propria indennità parlamentare,

Presidente, trovo di assoluta ragionevolezza l'emendamento 1.104, di cui è primo firmatario il senatore Centaro e assolutamente coerente poi con lo spirito della riforma che stiamo discutendo. Si sta introducendo il concorso di secondo grado, per cui si avverte l'esigenza che colui che accede alla magistratura abbia maturato altre esperienze di lavoro, sia dunque in grado di affrontare le responsabilità e l'impegno di una funzione così complessa forte di una esperienza che si è radicata in una serie di attività pregresse, di cui viene fatta espressa menzione, tutte attività naturalmente connesse. Trovo veramente singolare che, a fronte di questa esigenza di eterogeneità delle esperienze come prodromo dell'accesso in magistratura, non si voglia escludere tutta quella attività ulteriore che nell'ambito dell'amministrazione si sia realizzata, sia pure in contesti diversi. Trovo assolutamente irragionevole e confliggente con lo spirito della norma proprio l'impianto

queste considerazioni che tendono ad escludere che proprio l'esperienza e la maturazione possano essere condizione di apprezzamento ulteriore. Francamente resto assolutamente perplesso.

mi spiace che non sia presente il ministro Mastella, ma la stessa domanda potrei rivolgerla al sottosegretario Scotti, stante l'identica provenienza geografica. C'è una vecchia commedia di Eduardo De Filippo, «Natale in casa Cupiello», che aveva come *leitmotiv* il papà che chiedeva al figlio: «Peppiniè, ma ti piace 'o presepe»? E Peppiniello tutte le volte rispondeva

Ora, siccome, a differenza del Peppiniello di «Natale in casa Cupiello», immagino che non vi sia un conflitto generazionale figlio-padre, né - a dire la verità - riesco a intravedere un conflitto politico

a cercare di stimolare il relatore e, se del caso, anche il Governo a darci un minimo di motivazione rispetto a taluni

i docenti universitari potranno fare tranquillamente il concorso in magistratura, come già è previsto nell'emendamento che si vuole emendare. Qual è il problema? Davvero vorrei avere delle spiegazioni. Noi abbiamo una serie di categorie individuate come idonee a sostenere il concorso in magistratura. Due di queste escono positivamente dalle scuole di specializzazione, sia quelle per le professioni legali, sia quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 162. Un'altra categoria è quella degli avvocati,

*Rara avis*, insieme ad un'altra di cui all'emendamento successivo, è la categoria dei docenti. Che cosa si chiede di cambiare?

si richiedono cinque anni di servizio nei confronti di un funzionario dello Stato, che ha superato un concorso pubblico nella stragrande maggioranza dei casi con materie identiche a quello in magistratura, mentre i cinque anni non si richiedono per i docenti in materie giuridiche. Ma non solo.

di storia di diritto dell'Oriente mediterraneo o di filosofia del diritto, ossia sostanzialmente di tutte quelle materie che sono importantissime nella creazione della cultura di un giovane, ma che con il concorso in magistratura non c'entrano assolutamente nulla? Siccome credo che possiamo essere d'accordo in ordine al fatto che questa norma non sia sconvolgente sotto il profilo politico,

ai docenti in materie giuridiche, qualunque esse siano (anche quelle che con il concorso in magistratura non c'entrano assolutamente niente), che non fanno evidentemente concorsi simili a quello dei funzionari pubblici, non si richiede quel minimo di requisito di cinque anni. Vi dico un'altra cosa:

Probabilmente lo avete fatto perché ritenete non cumulabili gli anni, perché ritenete che l'esperienza in una determinata attività debba essere compiuta e sicuramente non è compiuta, secondo quella che è la vostra costruzione, una attività di due anni come funzionario dello Stato invece di cinque. E allora spiegatemi qual è l'esperienza che matura un docente in materie giuridiche il giorno dopo che ha vinto il relativo concorso e solo per questo può fare il concorso in magistratura senza quegli anni di fatica e di lavoro che vengono richiesti a tutte le altre categorie. Ove mai i colleghi, signor Presidente, volessero concedermi il supporto, chiedo il voto elettronico.

certo all'etnia del collega Palma, però credo che Luca Cupiello chiamasse il figlio Ninnillo, non Peppiniello: per la storia deve rimanere agli atti.

Senatore Castelli, vorrei farle notare innanzitutto che nella Conferenza dei Capigruppo nessuno, compreso lei, quindi, ha obiettato alla definizione del calendario che qui è stato proposto dal Presidente, che prevede la conclusione di questo provvedimento nella settimana in corso, cioè sino ad arrivare - lo ripeto per la terza volta - a sabato mattina. Dopo di che la Presidenza si è avvalsa del Regolamento del

ad armonizzare i tempi degli interventi con i termini del calendario». All'articolo 55, al comma 5, si dice, caro senatore Castelli, che «la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari determina di norma il tempo complessivo da riservare a ciascun Gruppo, stabilendo altresì la data entro cui gli argomenti iscritti nel calendario debbono essere posti in votazione». Di norma, quindi, noi stiamo già facendo un'eccezione, perché i tempi per ciascun Gruppo non sono stati definiti, ma è stato definito il tempo di conclusione del provvedimento. Pertanto, senatore Castelli, io non ho né usato violenza, né forzato il Regolamento, ma l'ho, al contrario, applicato alla lettera, rispettando alla lettera la decisione della Conferenza dei Capigruppo. Mi dispiace doverle rispondere in questi termini, ma questo è quello che ho fatto, rispettando peraltro le decisioni e le scelte di carattere politico che il Gruppo della Lega e i suoi singoli componenti intendono fare nel merito del provvedimento che stiamo discutendo e quindi votando, di conseguenza, rispetto a queste scelte. Senatore Galli, adesso può intervenire.

se mi concede una replica, perché la logica aristotelica vale per tutti. Lei mi conferma la giustezza dei miei ragionamenti, perché lo ha dichiarato lei che, di norma, i tempi vengono

È vero che abbiamo stabilito che si voterà entro sabato, per cui, se fosse sabato mattina, lei avrebbe tutte le ragioni per armonizzare i tempi; siccome siamo a martedì, credo che il nostro Gruppo abbia tutto il diritto di modulare i propri interventi come meglio crede, visto che siamo fuori dalla norma. Quindi, il fatto che lei cominci ad armonizzare il martedì, mi scusi, è eccessivo,

al che voteremmo il provvedimento domani sera e non sabato. Lei non può interferire sulle decisioni autonome di un Gruppo, su come noi vogliamo modulare gli interventi. La seconda questione che tengo a sottolineare

della situazione di non controllo di tutto quello che arriva da quel Paese dell'Estremo Oriente. È di questi giorni la notizia che ormai in molti Paesi indagini contro responsabili e funzionari di vari istituti europei, corrotti da aziende del Sud‑Est asiatico, dell'Estremo Oriente, interessate ad agevolare l'introduzione dei loro articoli nei nostri mercati,

se il Presidente mi dà un attimo di attenzione, non so se ha famiglia o altro, credo di sì; io ho dei bambini piccoli e mi dispiacerebbe che mettessero in bocca un dentifricio velenoso, perché è di questo che stiamo parlando - se qualcuno di quelli che va in Cina a stringere le mani insanguinate dei burocrati comunisti cinesi e che va a stipulare accordi per vendere quattro Ferrari o mettere quattro aziende di scarpe di Della Valle e compagnia, non ritenga di dover venire in questo luogo - visto che ne facciamo esplicita richiesta - a informarci

Napoli, Livorno, Trieste e Genova, dove arrivano i *container* dalla Cina, la Guardia di finanza non c'è. Tutte le volte che è stato effettuato un minimo di controllo, anche tramite Commissioni parlamentari, si è rilevato che i controlli sono

ma solo ieri reso noto. È stato inibito l'ingresso gratuito al Parco della Valle dei templi ad un gruppo di ragazzi di età inferiore ai 12 anni, che, pur cittadini italiani, avevano un requisito, non previsto dalle tariffe e neanche dalla circolare: avevano la pelle nera. Figli di immigrati, figli nati in Italia, cittadini italiani. Il consorzio che gestiva la biglietteria e che ha inibito l'ingresso al parco per voce del responsabile si è defilato da qualsiasi responsabilità, facendo riferimento ad una circolare regionale, che - a dire dell'assessore regionale ai beni culturali Lino Leanza - fa riferimento ad una burocrazia poco elastica, che è attiva in tutta Italia. L'interrogazione tende ad ottenere una risposta anche immediata alle dichiarazioni dell'assessore siciliano. Resta il fatto che il danno è stato fatto. È apprezzabile l'iniziativa del neosindaco di Agrigento, Marco Zambuto, che ha invitato i piccoli dell'associazione Ziggurat di Palermo (che opera nel quartiere multietnico Ballarò), garantendo loro la visita ai templi e la dovuta ospitalità.

riguardante la drammatica mancanza di personale all'INPS di Bolzano, che non può essere risolta, come in altre Province, con il trasferimento o la mobilità, sempre per le esigenze autonomistiche di bilinguismo.